Onorevoli colleghi, lo scorso 16 settembre è mancato il senatore a vita, Presidente emerito della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. La sua figura sarà solennemente commemorata dal Senato, alla presenza della famiglia, in una prossima seduta nella quale saranno ripercorsi i più significativi momenti della sua azione azione al servizio delle istituzioni repubblicane, sia nella veste di dirigente, Governatore della Banca d'Italia, sia come uomo di Governo e Capo dello Stato. Sono certo di manifestare i sentimenti di tutti voi nel rivolgere alla famiglia del presidente Ciampi, in particolare all'amatissima moglie, signora Franca, ai figli e ai nipoti, il cordoglio del Senato della Repubblica e la nostra affettuosa partecipazione al loro dolore e a quello di tutto il popolo italiano. Invito quindi l'Assemblea a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento in memoria del nostro illustre collega.

Grazie Presidente. ha avuto modo di evidenziare gli indiscutibili risultati ottenuti in questi due anni di Governo in un settore strategico, quello della giustizia, non soltanto per l'effettività della tutela dei diritti, ma anche in quanto fattore di sviluppo e di crescita.

Rendere la giustizia più efficiente e rispondente ai parametri del giusto processo in termini di tempi e di smaltimento di cause pendenti al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato e nelle sue istituzioni è una priorità. La percezione di affidabilità in termini di sicurezza, giustizia ed equità degli interventi costituiscono infatti il collante sociale di una comunità, quel vincolo di lealtà che si pone alla base di un positivo senso di appartenenza e di cittadinanza responsabile. Il disegno di legge n. 2067 rappresenta pertanto uno strumento di riforma in tale direzione e reca modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, nonché modifiche all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Una delle prime importanti problematiche che abbiamo dovuto affrontare in questa legislatura è stata infatti, in particolare, quella del sovraffollamento delle carceri, a cui ci aveva richiamato la Corte europea con la famosa sentenza Torreggiani, a seguito della quale lo stesso presidente della Repubblica, Napolitano, aveva chiesto l'impegno del Parlamento. Abbiamo trattato tale questione con responsabilità, senza ricorrere a strumenti straordinari, ma piuttosto l'abbiamo affrontata con interventi strutturali di modifica del sistema delle pene e delle misure di esecuzione delle condanne, con particolare riguardo alle misure alternative al carcere. misure che sono espressione di una concezione della funzione della pena in evoluzione, certamente attuativa del disposto costituzionale di cui all'articolo 27, che prevede una pluralità di pene che devono tendere alla rieducazione, alla risocializzazione e infine, pene riparative nei confronti della vittima e della società, senza rinunciare al principio della effettività e certezza della pena, andando a istituire la pena della detenzione domiciliare come pena principale e chiedendo che la detenzione in carcere costituisca in concreto l'*extrema ratio*, soprattutto in fase cautelare. Sono cosi diminuiti i ristretti negli istituti penitenziari e raddoppiati i condannati ammessi alle misure alternative, anche con l'istituto della messa alla prova per adulti. Registriamo oggi, pertanto, una riduzione delle presenze in carcere da 66.000 a 52.000 detenuti, su 48.000 posti, accanto ad un numero di detenuti in regime di esecuzione esterne al carcere, di quasi 40.000 unità, ma con una tendenza attuale, ahimè, ad un nuovo inizio di sovraffollamento per alcuni istituti. Tuttavia, i provvedimenti contenuti in oltre sei atti di Governo e Parlamento necessitavano di un riordino di sistema, coerente e strutturato. Per questo la delega contenuta nel disegno di legge n. 2067 rappresenta uno strumento necessario di riforma e di aggiornamento anche della fase dell'esecuzione penale con le modifiche all'ordinamento penitenziario. In tale quadro, l'articolo 31 del disegno di legge in esame introduce principi quali la semplificazione delle procedure per le decisioni della magistratura di sorveglianza, anche con l'implementazione del sistema della videoconferenza e del dibattimento a distanza, che, nella garanzia del diritto alla difesa, consentirebbe anche un significativo risparmio di risorse. richiede la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, in riferimento alla pena e ai presupposti soggettivi, eccetto per i reati più gravi quali reati di mafia e terrorismo. Il disegno di legge, inoltre, ribadisce la necessità di rafforzare quello che sin dall'inizio era il cardine del nuovo ordinamento penitenziario, ovvero l'obbligo dell'osservazione scientifica della personalità del condannato, al fine della individualizzazione del trattamento penitenziario, per un programma di reinserimento e recupero, che con l'offerta di diverse opportunità, tra formazione, istruzione e, soprattutto, lavoro,

La differenziazione del trattamento e il sistema regionale dei circuiti penitenziari, ancora in attesa di una completa attuazione, nonostante il seppur tardivo regolamento di attuazione dell'ordinamento penitenziario n. 230 del 2000, sono oggi ancor più necessari, con la nuova emergenza della radicalizzazione islamica in carcere, con quel proselitismo facilitato anche da modalità nuove di gestione dei detenuti, quali la sorveglianza dinamica a celle aperte in molti istituti. Fondamentali rimangono i principi ribaditi nella delega e consegnati al Governo, di valorizzazione del lavoro intramurario, ma anche all'esterno, ai come strumento di recupero sociale, in quanto elementi cardine del programma di trattamento penitenziario, in grado di riconnettere il condannato con il mondo esterno. Tuttavia, due questioni su cui richiama l'attenzione la delega sembrano rimanere ancora oggi in secondo piano, ovvero la questione del riordino della sanità e della medicina penitenziaria e il riconoscimento del diritto all'affettività relazionale con i familiari. Il carcere che si apre alla società esterna diventa permeabile e, grazie alla cooperazione con gli enti locali, l'associazionismo e il terzo settore, offre oggi opportunità di reinserimento sociale e occupazionale reali. Per questo è necessario potenziare l'organizzazione collegata all'esecuzione penale esterna sia in termini di compiti di sorveglianza per la polizia penitenziaria sia in termini di figure quali assistenti sociali, psicologi ed educatori.

il legislatore, al Capo IV - Disposizioni finali e transitorie - e segnatamente all'articolo 79, precisava che le disposizioni della legge si sarebbero applicate anche ai minori di anni diciotto fino a quando non si fosse provveduto con apposita legge. In questo modo riconosceva la necessità di una disciplina autonoma delle norme contenute nell'ordinamento penitenziario rivolte ai minori. Il riferimento non riguarda solo l'offerta di opportunità di istruzione, formazione e lavoro inframurario, ma riguarda anche i requisiti di ammissibilità delle misure alternative. In tale direzione occorre ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 125 del 25 marzo 1992, chiedeva al Parlamento una revisione dei criteri e dei limiti di ammissione alla semilibertà e all'affidamento in prova, al fine di distinguere la condizione del minore di età rispetto ai condannati adulti. Successivamente la stessa Corte con la sentenza n. 168 dell'aprile 1994, nel ribadire l'incostituzionalità di una pena per i minori che costituisca, di fatto, un ergastolo, imponeva «un mutamento di segno al principio rieducativo nei confronti di un soggetto che è ancora in formazione ed alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa», al fine di conseguire un efficace reinserimento sociale volto anche ad un pieno recupero finalizzato a scongiurare la recidiva a delinquere e una facile azione di proselitismo. occorre ricordare come la delega si inserisca in un contesto di accelerazione della costruzione di uno spazio di cooperazione giudiziaria comune europea, in attuazione del titolo V del Trattato europeo del 2009, per uno spazio unico di libertà, giustizia e sicurezza fondato sulla fiducia reciproca dei sistemi di giustizia nazionali e sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie anche attinenti all'esecuzione delle pene e delle misure alternative negli Stati membri diversi dallo Stato di emissione. lontani dalle regole minime per il trattamento dei detenuti risalenti al 1973, poi confermate dal Consiglio d'Europa nel 1987, la forte prospettiva di unione lanciata da ultimo dal Trattato di Lisbona del 2009, ai sensi dell'articolo 67, per un'effettiva cooperazione giudiziaria e di polizia. a partire dalla legge n. 354 del 1975, poi dalla legge Gozzini, con la quale sono state introdotte le misure alternative alla detenzione in carcere, e dalla legge Simeoni, con la quale si è evitato l'ingresso in carcere con la sospensione dell'ordine di esecuzione, tra passi indietro, quale la legge ex Cirielli e inasprimenti di vincoli, il nostro ordinamento oggi rilancia un modello di esecuzione penale segnatamente più moderno e volto al pieno recupero sociale del condannato, in linea con l'orientamento del sistema europeo

che ogni giorno vive nel carcere e ne subisce le sue permanenti carenze, in attesa di quel giusto riconoscimento, di quella valorizzazione che abbiamo promesso con la legge di stabilità di quest'anno e di quel riordino e riallineamento che lo equiparerebbero alle altre forze di polizia.

Prendiamo degli spunti, anche a caso, perché basta guardare qualsiasi norma per rendersi conto di come essa sia inconsistente, assolutamente inefficace o addirittura dannosa.

querela. Signori, in questa maniera andiamo a vanificare la possibilità di procedere nei confronti di moltissimi reati, perché a volte chi deve sporgere querela non lo fa magari per paura di una ritorsione, per dimenticanza, oppure perché particolarmente turbato dall'ipotesi di reato.

Ricordiamo anche tutte quelle ipotesi di violazione di domicilio. Ogni volta dovremo attendere che sia il privato a farsi carico dell'intera procedura per far andare avanti il processo.

possano leggere il contenuto dell'articolo che prevede la delega a rivedere l'ordinamento penitenziario. Si dice di favorire i trattamenti rieducativi, concedere benefici penitenziari per i condannati all'ergastolo,

Stiamo parlando della massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna. E poi, cos'è la sorveglianza dinamica?

quel ramo del Parlamento, che doveva avere la possibilità di andare avanti e diventare effettivamente legge. Si trattava di una norma sul giudizio abbreviato che escludeva la possibilità di ricorrere a questo istituto in alcune ipotesi, gravissime. Noi prevedevamo che non si potesse concedere la possibilità di ricorrere al giudizio abbreviato, ad esempio nel caso di sequestro di persona per scopi di terrorismo, per strage, per omicidio aggravato, per la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, il sequestro di persona a scopo di estorsione. Secondo noi il giudizio abbreviato, che prevede dei benefici di riduzione della pena, non deve essere concesso in queste ipotesi. In questo caso, il nostro emendamento, volto a introdurre tale previsione, è stato completamente dimenticato.

Noi non potremo mai approvare una riforma del processo penale finché restano in vita tutte queste misure. Dobbiamo eliminare la possibilità della custodia cautelare in carcere solo per i reati puniti fino a cinque anni. Vogliamo che sia eliminata la liberazione anticipata così come voi l'avete ampliata. Vogliamo evitare che vi siano ancora degli sconti di pena per le cosiddette condizioni inumane della detenzione. Vogliamo sia eliminato l'istituto della messa alla prova. Solo attraverso queste eliminazioni noi potremo arrivare ad approvare una riforma del processo penale. Ma soprattutto, e anche questa la consideriamo una lacuna gravissima, non si è parlato della legittima difesa.

Sono tutte ipotesi che non possono non essere valutate. Quindi, non possiamo fare una riforma del processo penale con delle mere limature.

fate finta di avere introdotto degli aumenti di pena seri nei confronti dei furti in appartamento e delle rapine, ma noi diciamo che così non va bene e proponiamo dei disegni di legge efficaci, perché solo in questo modo riusciremo ad avere un sistema penale serio.

già in sede di esame della questione pregiudiziale presentata dal senatore Caliendo avevo fatto delle osservazioni in ordine ai profili di incostituzionalità del disegno di legge

normativa, ovvero alternare a breve distanza di tempo interventi di segno diametralmente opposto, in genere per assecondare le presunte volontà Si parla anche di pendolo legislativo per rappresentare efficacemente la continua oscillazione delle leggi da un estremo all'altro. Nel disegno di legge che oggi oggi esaminiamo vi è qualcosa di più di questa schizofrenia legislativa: un qualcosa di sconcertante,

collega Barani - in un paziente psicotico affetto da personalità multiple, idee e visioni del diritto penale, della sanzione e del processo diametralmente opposte.

Si vanifica l'effetto di questo innalzamento di pena - da qui la schizofrenia - perché all'articolo 36

la pena massima per la quale poteva chiedere la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena era di tre anni. Ora è stata portata a quattro anni: ditemi voi se per un furto in appartamento

di un condannato di vedere sospesa l'esecuzione della pena comminatagli, risponde magari rigettandola dopo quattro anni. Quel signore, che ha consumato il reato di furto in appartamento, avrà quattro anni di tempo per accumulare eventualmente altre condotte illecite, quindi consumare altri reati di questo genere. Vi è poi il sistema delle deleghe. Signori, queste sono deleghe in bianco; noi diamo

determinati requisiti. Se leggete le deleghe inserite in questo disegno di legge vi accorgerete che in sostanza si tratta di deleghe in bianco. Quindi, non sappiamo

Il senatore Casson, relatore del provvedimento, in un primo momento aveva immaginato

della prescrizione per le sentenze di condanna. Noi non siamo contrari a vedere ulteriormente allungato il termine della prescrizione;

ho visto che l'ipotesi della sospensione o dell'interruzione dell'azione giudiziaria promossa dallo Stato quando la durata del processo va oltre certi limiti

"prescrizione del reato": se un fatto si è commesso o comunque c'è stato non si prescrive affatto; diciamo che si prescrive la titolarità dello Stato a perseguire quel determinato soggetto per quel determinato reato.

anche nel rispetto dell'articolo 111 della Costituzione, in particolare per il reato di corruzione, che per quanto mi riguarda è un reato odioso

incide ancora più fortemente sotto il profilo culturale dei rapporti tra cittadino e istituzioni, perde la fiducia nei confronti delle istituzioni

avevo altresì immaginato di svuotare un po' questo paniere, perché se inseriamo molti reati in questo paniere si vanifica l'effetto. Non si è potuto dire di no; il mio emendamento è stato accolto in Commissione: come si faceva, infatti, a negare che questo tipo di reato dovesse avere una una corsia preferenziale in un momento in cui si avverte, da parte dell'opinione pubblica, la gravità di questi fatti? Tuttavia ho fatto questo immaginando di equilibrare

perché non vi era accordo; alla fine si è giunti a questa soluzione povera, che consiste nel ridurre a un anno e sei mesi la sospensione dopo la sentenza. Insomma, un'accozzaglia di norme che non stanno insieme, neanche sotto il profilo dell'armonia normativa. Noi tra poco faremo le dichiarazioni di voto, se ci sarà concesso, visto che si parla di fiducia; non so, queste sono valutazioni che fa il Governo con la sua maggioranza.

Non votando la fiducia dimostriamo che noi, sui singoli provvedimenti, liberamente, senza avere condizionamenti di sorta, decidiamo se votarli o meno. Ripeto, se viene posta la fiducia su questo provvedimento io personalmente non la voterò mai, perché non posso essere accomunato a quel legislatore schizofrenico di cui vi ho illustrato il tratto poc'anzi.

danni contro il patrimonio, reati di tipo predatorio, che si accompagnano, sempre più spesso, ad efferata violenza nei confronti delle persone, sia che si tratti di episodi di furto in strada o in abitazione, sia rapine in esercizi commerciali e in attività professionali. Tutto questo avviene nel momento in cui il Paese attraversa ‑ lo sappiamo ‑ una crisi sociale che non ha precedenti, vuoi per problemi economici, vuoi anche per una presenza così numerosa e quasi fuori controllo, ormai, sul nostro territorio di persone provenienti da altri Paesi, extracomunitarie, che spesso non risultano

esistono clandestini non identificati che si danno anche alla vita criminale. Le cronache ci raccontano vari episodi; l'ennesimo è accaduto l'altro ieri nella mia città, Verona, in cui un pluripregiudicato clandestino, che già aveva ricevuto un

una volta catturato è stato condotto in carcere, giudicato per direttissima e il giorno dopo scarcerato, nonostante i precedenti penali e nonostante il provvedimento di espulsione non eseguito. Chiaramente la vittima del reato al pari di tutti noi e di tutti i nostri concittadini - di fronte a episodi come questo rimane totalmente sconcertata e si chiede dove sia la risposta della giustizia, dove siano la certezza del diritto e, soprattutto, la certezza della pena. È stato scarcerato perché il giudice, in quel caso, ha ritenuto che delle circostanze attenuanti o una particolare ricostruzione dei fatti non comportassero la comminazione di una pena tale da condurre questa figura

comporta degli episodi di questo tipo. Una persona che commette un reato, che viene percepito come un reato di grande pericolosità sociale da chi lo subisce e dalla comunità intera, viene scarcerata perché magari le prove, le ricostruzioni la norma vengono interpretate in un modo diverso da quello che avrebbe potuto fare un altro giudice. Il riscontro però è sempre che chi commette un reato, un criminale, per andare davvero in galera, per andare davvero in carcere nel nostro Paese, chissà cosa deve fare. Questo non è più tollerabile. La domanda di sicurezza dei nostri cittadini nasce dall'emergenza e dal fatto che si sentono non tutelati e abbandonati dallo Stato, che non sa dare una risposta di fermezza e di rigore. Perché ho fatto questa premessa? Vorrei rivolgere un richiamo forte al Governo, alla maggioranza e a tutte le forze di opposizione, che hanno il compito di cercare di portare a termine al meglio delle modifiche normative in un settore così importante e vitale per il Paese.

(furti e rapine), segua una pena esemplare, che venga inflitta e che venga espiata per davvero, fino alla fine. Abbiamo l'occasione di intervenire subito per dare questa risposta di giustizia ai nostri cittadini,

pagherà per quello che ha fatto, rimanendo in carcere. Il problema delle presenze in carcere dei detenuti, del sovraffollamento e quant'altro lo affronteremo e lo dovremo affrontare in molti altri modi, ma certamente non con il buonismo

soprattutto quando un criminale entra nella dimora privata di qualcuno, all'improvviso (magari di notte), o nell'ambito della sua attività (di un negozio o di un'attività professionale), compromettono la sicurezza non soltanto della vittima che subisce il reato, ma - ripeto - di un'intera comunità. Faccio anche presente a Governo e maggioranza che l'occasione è quella di ridisegnare le norme in modo puntuale e preciso.

che prevede una norma di facile interpretazione e soprattutto di facile applicazione: una pena secca, molto più alta (triplicata), senza possibilità che vengano concessi sconti, benefici o misure premiali e senza la possibilità che le attenuanti prevalgano sulle circostanze aggravanti (sempre nei casi di furti e rapine), senza la possibilità che siano concessi degli sconti o anche la misura degli arresti domiciliari o l'applicazione del fatto di lieve entità. Perché lo dico e perché è possibile farlo? Se noi paragoniamo il nostro ordinamento a quello di altri Paesi (non mi riferisco alla solita Germania, ma penso alla stessa Romania), notiamo che questi hanno un sistema penale che, per il furto e la rapina, prevede delle pene che sono molto più alte delle nostre. Il nostro Paese, rispetto a chi viene da altrove da noi, dà l'immagine di un Paese talmente buonista, talmente privo di rigore e di fermezza, da far pensare quasi al paese di Bengodi, in cui uno arriva e può delinquere indisturbato, perché tanto sa che rimarrà Non soltanto alcuni Stati europei (ma se guardiamo anche altrove in Occidente) prevedono pene più alte, ma prevedono pene secche in modo che non vi siano possibilità di interpretazioni fuorvianti. Abbiamo presentato anche emendamenti specifici che vanno in questa direzione. direzione. Colleghi, lo dico soprattutto al Governo e alle forze di maggioranza, ma anche ai colleghi degli altri partiti di opposizione: abbiamo la possibilità di congegnare un sistema efficace, rigoroso e preciso che finalmente porti questo ordinamento verso la direzione della certezza della pena per dare una per dare una risposta di sicurezza ai nostri cittadini ed è questo ciò che ci chiedono. Non ci chiedono di argomentare tanto sulla prescrizione; a loro questo sì interessa, ma interessa fino a un certo punto. Vogliono una risposta di sicurezza rispetto a quanto quotidianamente vedono e soprattutto vivono sulla loro pelle, nelle loro case e nelle loro attività. Con i nostri emendamenti questo si può fare. E quindi auspico che vi sia innanzitutto la volontà

Signor Presidente, il disegno di legge che oggi esaminiamo è complesso, corposo e tratta una materia estremamente delicata. Ci sarebbe da discutere per mesi vista l'estensione e l'importanza delle modifiche che si vogliono apportare all'ordinamento penale. vorrei ripercorrere alcuni punti imprescindibili del provvedimento. Tra l'altro devo aggiungere che il provvedimento, così come è arrivato in Aula, manifesta dal mio punto di vista (evidentemente non intendo impegnare il Gruppo al quale appartengo) ancora

tenga conto del fatto che c'è, anche nell'ambito di alcuni settori della maggioranza, uno stato di disagio e di perplessità su alcuni punti specifici. dobbiamo ripercorrere alcuni punti. Tra i 40 articoli ci sono alcuni punti che riguardano la riforma della prescrizione, l'inasprimento delle sanzioni per i reati gravi e odiosi, come lo scambio elettorale politico‑mafioso, il furto e la rapina, la rapina, che possiamo anche apprezzare positivamente. Vengono dettate norme di semplificazione del processo penale. Vengono assegnate deleghe al Governo per il riordino della delicatissima materia delle intercettazioni e per l'altrettanto fondamentale riforma dell'ordinamento penitenziario. Al riguardo, auspichiamo che il Governo faccia buon uso di queste deleghe: mi riferisco in particolare all'argomento che riguarda le intercettazioni

Non viene nemmeno trascurato nel provvedimento il capitolo della semplificazione delle procedure in materia penale a cui è dedicato il titolo del disegno di legge. Sul tema della prescrizione la decisione di sospendere di un anno e sei mesi il decorso della prescrizione dopo il primo grado e altrettanto dopo l'appello soddisfa l'esigenza processuale di termini più lunghi per il giudizio, anche se personalmente, a dire la verità, ho sempre auspicato esattamente il contrario, che il giudizio avvenga in tempi ragionevoli, anche perché ricordiamo che siamo sempre vincolati al criterio fondamentale che è quello della giusta durata del giudizio. potrebbero dilatare enormemente i tempi del giudizio e non vorremmo che questo provvedimento determini effetti di questo genere. Essi rappresentano, infatti, al di là degli esiti del giudizio stesso, comunque già di per sé

il regime della prescrizione, alla fine del lavoro della Commissione, in alcuni punti è rimasto di stampo liberale e quindi abbastanza equilibrato, come previsto dal codice del 1930, seppure questi correttivi che determinano l'aumento dei termini, come dicevo poc'anzi, per le fasi di impugnazione, sia in appello sia in Cassazione, garantendo in ogni caso l'esaustivo del rispetto del principio della ragionevole durata del processo, di fatto, a mio avviso presentano delle criticità. Per quanto riguarda la delega in materia di intercettazioni, voglio sottolineare il rilievo attribuito al principio della garanzia della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche intercettate, in conformità all'articolo 15 della Costituzione. Da questo punto di vista sembra assolutamente positiva l'attenzione alla tutela delle intercettazioni a carico delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, anche rispetto alle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini della giustizia penale. Sarà punito anche chi diffonderà intercettazioni illegali per danneggiare la reputazione altrui. Infine, la Commissione ha avuto il merito di dettare criteri direttivi precisi e puntuali relativi alle intercettazioni con i captatori informatici, i cosiddetti virus *trojan*. Di primario rilievo appaiono anche alcuni profili della delega di riforma dell'ordinamento penitenziario: mi riferisco all'accesso alle misure alternative ai benefici penitenziari, di cui si intende facilitare l'utilizzabilità, all'individuazione di attività di giustizia riparativa, all'incremento e alla valorizzazione delle opportunità di lavoro e volontariato per i detenuti, tutte intese come momenti qualificanti del percorso di recupero sociale degli stessi. Positivo è anche il rilievo attribuito alle esigenze educative dei detenuti minorenni, agli specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri. Il lavoro è stato intenso, ci sono stati dei momenti di vivo confronto tra le varie anime politiche della maggioranza e anche tra maggioranza e opposizione. La discussione ha rappresentato un' occasione per raggiungere diversi punti di intesa, peraltro più alti rispetto alle posizioni di partenza, trovando delle soluzioni condivise. Per concludere, il testo del disegno di legge all'esame, come modificato approfonditamente dalla Commissione giustizia, è stato favorevolmente accolto dal Consiglio superiore della fatto questo non unico, ma certamente raro rispetto a quanto accade o è accaduto normalmente, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza. Quindi, credo che nel complesso possiamo manifestare una certa soddisfazione e colgo l'occasione per ringraziare, oltre ai membri della Commissione, il Presidente della Commissione giustizia, il senatore D'Ascola, per la magistrale gestione

sollecito nuovamente l'attenzione del Governo per una più attenta valutazione del testo che, in caso di eventuale richiesta di voto di fiducia, verrà portato all'attenzione e all'apprezzamento dell'Assemblea e, soprattutto, della maggioranza.

da un mancato contrasto alla corruzione e quindi dalla prescrizione, che fa decadere i processi. Questa anomalia del nostro sistema viene sottolineata anche dall'OCSE e dalla Corte di giustizia europea, ma, come ben sappiamo, ci facciamo imporre dall'Europa solo le cose che, in qualche misura, ci convengono e quando, invece, è il caso di dare corso a dei giusti provvedimenti, non lo sappiamo o non lo vogliamo fare.

la sua differenza, ma non basta. Sappiamo che c'è bisogno di fare la differenza affinché non si verifichino più prescrizioni come quelle di Porto Marghera, del caso Eternit, del processo Cassiopea, della discarica di Pitelli, del processo Artemide

ci sono solo i reati ambientali; quanto ci costa la corruzione? Non certo 60 miliardi, che sembra una cifra falsa. Forse ce ne costa 100 miliardi. La verità è che non si sa quanto. Quello che si sa per certo è che la spesa per contratti, opere, forniture e servizi servizi pubblici è del 40 per cento in più per la corruzione. Questo è un dato della Corte dei conti. È un dato sicuramente certo.

Questa è l'Italia che vogliamo, visto che ancora oggi non stiamo risolvendo il problema? Certo, la prescrizione nasce per dei motivi molto ragionevoli: avere un sistema economicamente sostenibile,

15 giudici per ogni 100.000 abitanti, contro una media che va dai 25 fino ai 60 giudici per 100.000 abitanti e abbiamo una mancanza strutturale dell'organico di oltre il 26

Signor Presidente, onorevoli senatori, la proposta di legge di riforma del processo penale, pur costituendo un passo in avanti, non prefigura una soluzione di cambiamento radicale della disciplina della prescrizione, così come ci si sarebbe aspettati e come da anni chiedono a gran voce tutti gli osservatori, da Caselli a Gratteri, da Roberti a Cantone, da Davigo, da Libera a Riparte il futuro. non basta allungare solo un po' i tempi della prescrizione tra appello e Cassazione se il nostro Paese intende lasciarsi definitivamente alle spalle il dato dei circa 150.000 processi all'anno che vanno al macero. Eppure l'Italia è uno dei Paesi con il più alto indice di percezione della corruzione in Europa e sappiamo benissimo che la grande insidia tipica delle pratiche corruttive, rappresentata dagli accordi occulti tra corrotto e corruttore in assenza di denunce,

Si tratta della famigerata cosiddetta legge ex Cirielli del 2005, che ha prodotto effetti devastanti sul sistema processuale. Prima del 2005 il termine di prescrizione per un reato di corruzione era di quindici anni, ma dopo il 2005 è stato ridotto a sette anni e sei mesi fino alla riforma del 2012. Sui processi coinvolti dalla prescrizione per reati particolarmente gravi, come i delitti causati da incidenti sui luoghi di lavoro, nonché i delitti ambientali e quelli relativi all'amianto, gli emendamenti che ho presentato vanno nella direzione già illustrata dal senatore Casson. Si tratta di situazioni particolarmente odiose. Ricordo a me stessa che sono andati prescritti i reati del G8 di Genova, dove inermi manifestanti sono stati sorpresi nella notte nella scuola Diaz e picchiati selvaggiamente, come ha riconosciuto una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo cosiddetta sentenza Cestaro del 2015). Sono andati prescritti i reati dei vertici dell'Eternit per le morti da amianto e rischiano di andare prescritti i reati dei dirigenti delle Ferrovie dello Stato italiane per l'immane strage di Viareggio. Se aboliamo l'articolo 161, comma 2, si coglie anche meglio il senso del mio secondo emendamento, volto a introdurre, tra le cause interruttive della prescrizione, la sentenza di condanna di primo grado. Al momento, nell'articolo 160 il rinvio a giudizio interrompe la prescrizione, pur se l'effetto di tale interruzione è sterilizzato dalla cosiddetta Aggiungere la condanna in primo grado come fatto interruttivo (e non sospensivo, come proposto nel testo) sarebbe più coerente, in quanto il nostro ordinamento si collocherebbe così sulla scia delle maggiori democrazie europee. Del resto, in Germania un reato grave, con una pena compresa tra i cinque e i dieci anni (cioè la nostra corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio), si estingue per prescrizione in dieci anni. se si verifica l'interruzione, si arriva fino a vent'anni, cioè il doppio del termine legale di prescrizione. In conclusione, avrei auspicato su questo singolo punto un approccio più deciso. più deciso. È assolutamente evidente che una riforma più incisiva del regime della prescrizione non solo migliora il nostro sistema della giustizia, ma può avere effetti decisivi nell'impatto sull'economia italiana e nel contrasto dei suoi mali endemici. Infatti, la corruzione, come ci ha ricordato più volte la Corte dei conti, non solo riduce la qualità dei servizi incidendo sulle entrate fiscali, ma aumenta anche l'ingiustizia sociale e la povertà.

all'inizio del suo intervento la collega Stefani ha parlato di una occasione persa. Ed è proprio questa la sensazione che tutto il Gruppo della Lega Nord ha nei confronti di questo provvedimento. Era un provvedimento che doveva dare risposta a una delle vere emergenze del nostro Paese, cioè l'esigenza dei nostri concittadini di sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni e nelle proprie città rispetto ad episodi di criminalità che sono ormai sempre più diffusi e finiscono, immancabilmente, con la liberazione anche di quei pochi delinquenti che vengono arrestati. Ciò non avviene perché non vi sia la possibilità di combattere questi fenomeni o non vi sia la possibilità di mantenere in carcere coloro che commettono questi reati; questa situazione esiste nel nostre Paese è perché c'è una espressa volontà, da parte di questa maggioranza, di non assicurare alle patrie galere coloro che commettono questi reati. E lo possiamo dimostrare con i fatti, con tutti quei provvedimenti che, durante questa legislatura, questa maggioranza ha approvato a tutela dei delinquenti e contro la sicurezza dei cittadini. Il decreto legislativo del 16 marzo 2015, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolari reati considerati di di scarso impatto sui cittadini, è stato approvato da questa maggioranza e non certo ereditato da situazioni precedenti e da vecchie legislazioni. Così anche il decreto-legge del 1° luglio 2013, che prevede una custodia cautelare più bassa,

Gruppo LN-Aut)*. Voi siete complici di questa situazione aberrante e siete complici dei delinquenti che ogni giorno fanno violenza contro i nostri cittadini. A testimonianza di quanto affermo io vi riporto due degli infiniti casi che avvengono tutti i giorni sul nostro territorio. È notizia della settimana scorsa l'arresto di due cittadini extracomunitari di origine marocchina

per costringerla a dare informazioni rispetto ai soldi che teneva in casa. Ebbene, questi due cittadini marocchini sono irregolari, quindi, non dovevano essere presenti nel nostro Paese e, avendo già vari precedenti penali, dovevano essere in carcere per reati già commessi. Invece, grazie alla legislazione approvata da questo Parlamento, da questa maggioranza, quei due cittadini marocchini hanno potuto fare altre vittime. risalente alla settimana scorsa, riguarda un cittadino di Legnaro, in provincia di Padova, sempre in Veneto. Walter Onichini è stato accusato,

mentre il cittadino albanese, di ventiquattro anni, ladro, che voleva derubarlo e voleva dunque commettere un reato, ha addirittura chiesto un risarcimento di 300.000 euro. Questo è il quadro più evidente di ciò che è ciò che è l'Italia. Il Bengodi della criminalità, il luogo dove coloro che sono dediti a queste attività hanno la certezza di poter fare ciò che vogliono e lo fanno. E lo fanno, non perché la politica sia tutta uguale o perché non ci sia la possibilità di dare risposte a questa emergenza, ma perché si trova in una situazione favorevole in cui maggioranza e Governo non hanno a cuore la sicurezza dei cittadini, ma continuano a varare provvedimenti che non garantiscono sicurezza, ma esclusivamente l'impunità di coloro che delinquono e che ogni giorno rendono le nostre città insicure.

non posso aggiungere granché a quanto il mio collega Falanga ha poc'anzi detto in quest'Aula. può svolgere la funzione di giurista, può svolgere quella di filosofo vorrei allora domandare agli illustri relatori

e alle libertà dei cittadini, e cioè quel diritto negativo cui Isaiah Berlin faceva riferimento quando parlava di diritti inalienabili di cui il cittadino è portatore e che non sono nella disponibilità di alcuna autorità. Più alto è il tasso di questi diritti, più libero e garantito è il cittadino all'interno dello Stato. Voi, sostanzialmente, pur avendo da modificare e registrare tutta una serie di questioni, sostanzialmente arrabattate una serie di norme e ve ne approfittate, per non disturbare le anime ben nate dei magistrati, magistrati, compresa una norma che consente loro di fare le sentenze con maggiore calma e di celebrare i processi con maggiore tranquillità. Partiamo, cioè, dall'efficientamento della giustizia, scriviamo sul frontespizio di questo provvedimento che è volto a ottenere

Ora, io vorrei dire ai colleghi e ai dotti giuristi: ma del reato di concorso esterno che non è tipizzato, che consente a taluni pubblici ministeri di fare uso e abuso, sia della direzione distrettuale antimafia che della magistratura ordinaria, quando ne vogliamo parlare? Quando vogliamo parlare della carcerazione preventiva, che è diventata l'anticipazione di una pena, ben sapendo che quel processo non si celebrerà o, se arriverà alla fine, dopo decenni - in questo caso dopo un ventennio sarà del tutto ininfluente e anacronistico rispetto sia alla riabilitazione di colui che è stato assolto, sia al contesto politico, sociale e amministrativo all'interno del quale si è voluto incidere? Quindi noi saremo un popolo di inquisiti. Saremo un popolo che, assunta un'ipotesi di reato, una delazione, fosse anche un'antipatia - molte volte è questione di simpatia e di antipatia, perché non si riesce a capire come mai si colpisca uno e non un altro che pure si trova nella stessa condizione

che ne determini la condanna o l'assoluzione. Sembra che voi viviate in un contesto lunare, come se questa non fosse l'epoca in cui i processi si celebrano sui giornali, nei *talk show*; l'epoca in cui i magistrati non parlano più per sentenze, ma fanno le conferenze stampa il giorno successivo a quello in cui hanno emesso provvedimenti restrittivi, ammannendo alla stampa per vere e certe le tesi accusatorie,

con tutto il rispetto che le è dovuto. Invece di porci il problema di velocizzare la giustizia e di imporlo ai magistrati, ovviamente fornendone gli strumenti - mi sembra di aver ricordato che questo Governo voleva stanziare un miliardo per la giustizia qualche tempo fa - che cosa facciamo invece? Creiamo l'ulteriore comodità, a chi si inquisisce prima e a chi si giudica dopo, di poterlo fare, per alcuni reati contro la pubblica amministrazione,

il numero dei processi andati in prescrizione si è dimezzato - questo lo dice la statistica e non io, che non sono un tifoso della Cirielli - in questa veste mi sia consentito con grande umiltà

dalla disaffezione e dalla sfiducia che in certi contesti si aveva verso lo Stato e la sua capacità di fare giustizia,

perché va nel senso contrario a quella rapidità, a quel sentimento di giusta giustizia - consentitemi di usare questo pleonasmo al quale tutti gli uomini aspirano, perché non fa carico ai magistrati di accelerare le procedure e non si pone il problema che esiste un mare tra l'indagato e il condannato. Un'altra delle follie di questi mesi è la scemenza, che alcuni vanno accreditando a ogni piè sospinto, che possa esistere un'etica che viene prima di quella contenuta nella legge.

la morale o il concetto morale di qualcuno che ritiene debba essere anteposta a quella prevista dalla legge. Se passa l'idea che tutti gli indagati sono colpevoli apoditticamente o sono indegni di ricoprire cariche o di candidarsi - ne abbiamo viste e sentite di tutti i colori - allungando i termini della prescrizione, state sostanzialmente dando una mano a chi vuole instaurare in Italia questo metodo sbrigativo di giustizia politica, perché non si può definire diversamente. Allora, con buona pace di tutti quanti, esorto i dotti colleghi a porsi il problema della tipizzazione del reato di concorso esterno - noi vorremmo sapere cosa

Possiamo sottrarre il cittadino alle angherie e alle approssimazioni di chi lo indaga? Questo è tutto.

essenzialmente la capacità di limitare l'arbitrio dello Stato, di ogni forma di potere,

Noi siamo un'Assemblea elettiva che rappresenta la Nazione e deve rappresentare innanzitutto la difesa dei valori fondanti della Repubblica, che sono i diritti e le libertà dei suoi cittadini. E questa legge non li tutela: aggrava la situazione, piega le libertà e i diritti dei cittadini a maggior abuso e a maggior arbitrio da parte dello Stato.

in discussione è estremamente significativo, molto ampio nella portata per la giustizia penale e contiene un provvedimento sul quale mi soffermerò. Mi concentrerò soltanto sul primo comma dell'articolo 12, sul principio di delega che porta la lettera *d)*, che riguarda il problema delle persone con disturbo mentale soggette a provvedimenti da parte della giustizia.

Se tale principio dovesse rimanere così come è, farebbe fare un tremendo passo indietro alla situazione delle carceri e delle persone con disturbo mentale, riprendendo i principi

le persone che sono in attesa di accertamento della proprie condizione di salute mentale, oppure coloro che sono imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, oppure persone condannate che hanno visto ingenerare in loro problemi di salute mentale dopo la carcerazione e, quindi, durante la detenzione. Questi erano proprio i casi per i quali avevamo

ovvero che fosse attivata la rete delle strutture, dentro e fuori le carceri, che si occupano a pieno titolo dei problemi della salute mentale dei detenuti, degli imputati e di coloro che hanno bisogno di un accertamento della loro situazione mentale.

siano istituite le sezioni psichiatriche, con articolazioni specifiche; che vi sia l'osservazione psichiatrica, ovvero che siano garantiti ai detenuti ai quali sono sopraggiunti problemi di disagio mentale tutti i trattamenti psicologici, psicosociali e sanitari necessari per il loro e la loro riabilitazione, per quanto possibile; e, soprattutto, che gli istituti penitenziari si raccordino con i servizi sanitari delle aziende sanitarie competenti e delle Regioni affinché questo avvenga in presenza di una dotazione di personale specializzato adeguata per rispondere ai bisogni della popolazione carceraria che presenta problemi di salute mentale.

siano ricoverati nelle residenze (REMS) prosciolti e condannati, imputati e persone solo in attesa di accertamento delle loro condizioni di salute mentale:

avevamo superato, prevedendo che la tutela della salute delle persone in carcere fosse adeguata, al pari di quanto succede per le persone che non sono private della loro libertà.

che prevede, appunto, che le aziende sanitarie, le Regioni e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria lavorino per garantire la tutela della salute delle persone con disturbi mentali, così come previsto dalla normativa.

Sappiamo che, rispetto all'emendamento che abbiamo presentato, hanno proposto una modifica che condividiamo pienamente e che, anzi, è ancora più chiara rispetto a quanto abbiamo scritto. Riteniamo che questo emendamento sia fondamentale per evitare che il Paese faccia un passo indietro di dieci anni nella tutela della salute

che può apparire piccolo e di scarso rilievo rispetto alle dimensioni del provvedimento, ma che, per soggetti particolarmente fragili, è fondamentale, soprattutto perché conferma che le amministrazioni regionali e centrali devono fare ciò che la legge chiede loro di fare. Tutte le volte che non lo fanno - purtroppo, qualche volta, Regioni, ASL e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non hanno messo in atto i provvedimenti che sarebbero necessari - non possiamo, solo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, non ci piace questa riforma, per motivi di merito e di metodo. Rispetto al metodo seguito, ricordo che la proposta di legge in discussione prende le mosse da un disegno di legge presentato dal ministro della giustizia Orlando, di concerto con i ministri Alfano e Padoan, che in buona parte assume la forma di delega al Governo. E qui, signor Presidente, siamo veramente al paradosso. Non è accettabile che una norma che interviene, tra l'altro, per modificare la delicatissima disciplina delle intercettazioni non sia fatta dal Parlamento. Non è accettabile che sia sottratto ai cittadini un dibattito parlamentare partecipato, pubblico e trasparente. Non è accettabile che questa norma venga redatta nel segreto di qualche ufficio ministeriale - speriamo almeno che sia ministeriale magari avvalendosi dei consigli e delle consulenze di nuovi rappresentanti della maggioranza come Denis Verdini che, in materia di intercettazioni, potrebbero certo avere una certa competenza, ma non altrettanta garanzia di agire nell'interesse pubblico. Ma, al di là della scelta inopportuna della delega, è di tutta evidenza che la legge delega deve essere o dovrebbe quanto meno essere di origine parlamentare e non certo governativa, perché con la delega il Parlamento pone dei paletti che il Governo deve rispettare. Ma, siccome in questo caso la delega è di iniziativa dello stesso Ministro della giustizia, allora siamo al paradosso dei paradossi: il paradosso di un Governo che delega se stesso a disciplinare una materia delicata come quella delle intercettazioni secondo criteri e paletti paletti posti dal Governo stesso. E magari ci metterà pure la fiducia, per evitare la pur minima modifica parlamentare e la pur minima discussione sugli emendamenti. Ma allora, signor Presidente, qual è il ruolo del Parlamento? Qual è il ruolo di questo Senato? Cosa stiamo a fare qui? Stiamo forse a ratificare decisioni prese altrove? Sembra che quella cui stiamo assistendo sia una vera e propria anteprima di quanto succederà poi abitualmente, ogni giorno di legislatura, con la riforma costituzionale Boschi-Renzi-Verdini. Avremo, cioè, un Parlamento umiliato, ombra di se stesso, ridotto al ruolo di ratificatore di decisioni prese chissà dove (ovviamente non in Parlamento). Insomma, se nel metodo questo provvedimento è inaccettabile, nel merito per taluni versi è anche peggiore. Mi soffermo in particolar modo sulle intercettazioni. Innanzitutto questa riforma attribuisce al Governo una delega eccessiva, sostanzialmente una delega in bianco, giustificata con l'esigenza di tutela della *privacy* dei cittadini. Poco importa che in Italia non vi sia un solo cittadino su 60 milioni (che non sia un politico) che si lamenti della presunta invasione della riservatezza. Peraltro, guardando al *database* del Garante per la protezione della *privacy*, troviamo che i casi acclarati di effettiva violazione di *privacy* sono stati dodici in venti anni: nulla di nulla. luogo, e come se non bastasse, i magistrati non saranno più liberi di utilizzare i *software* che ritengono più idonei per effettuare le intercettazioni. Dovranno limitarsi all'utilizzo di quelli certificati da un organo politico, e cioè dal Ministero della giustizia. In altre parole, sarà il Ministro a comunicare ogni anno l'applicazione informatica che dovrà essere utilizzata, dando così modo a delinquenti, corrotti e corruttori di dotarsi delle giuste e corrette e corrette contromisure, in grado di annullare l'effetto delle indagini a loro carico. In terzo luogo, non potranno più essere intercettati quei criminali che organizzano - ad esempio una cena a casa propria, per parlare di mazzette, appalti, voto di scambio, eccetera, sempre che il magistrato non abbia la certezza che in quel luogo si stiano compiendo attività criminose. Se in altre parole fino ad oggi il magistrato può ricorrere all'uso delle intercettazioni se ritiene fondatamente che si stia compiendo un crimine, in futuro occorrerà che ne abbia la certezza. E questo è gravissimo, perché presuppone la flagranza del reato e, quindi, esclude questo strumento nella stragrande maggioranza dei casi. In quarto luogo, il disegno di legge prevede il carcere prevede il carcere addirittura fino a quattro anni per tutti coloro - giornalisti esclusi - che diffondono riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, eseguite «fraudolentemente» e suscettibili di causare un danno d'immagine al soggetto registrato. Questa norma rappresenta un potenziale bavaglio per tutti i cittadini, per tutti coloro che non potranno più compiere registrazioni di incontri, riunioni o consigli comunali, considerato che dalla diffusione delle registrazioni potrebbero poi doverne rispondere penalmente. L'avverbio «fraudolentemente», infatti, è troppo generico e fonte di grandissima incertezza. Solleverà inevitabili dubbi sia interpretativi che applicativi. In quinto rischiano di non essere più consentite la divulgazione e la pubblicazione di risultati di intercettazioni che coinvolgono soggetti pubblici, Ministri, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci

sono tutti scandali che hanno portato alle dimissioni di Ministri della Repubblica che probabilmente non sarebbero mai emersi. Eppure non è solo il Movimento 5 Stelle a nutrire pesanti riserve rispetto a questa riforma: il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Piercamillo Davigo, si è detto contrario, come il suo predecessore Rodolfo Sabelli. L'ANM ha dichiarato che «una delega siffatta rischia di trasformare il legislatore delegato» - il Governo - «in legislatore ordinario» ha rilevato che la delega contenuta nel disegno di legge sulla riforma del processo penale «presenta aspetti problematici per il suo carattere generico». E si capisce bene il perché: è sostanzialmente una delega in bianco. Un senatore di maggioranza in Commissione giustizia l'ha definita «incostituzionale» per lo stesso motivo. Anche i procuratori capo delle maggiori città italiane, auditi in Commissione, si sono dichiarati unanimemente contrari a un intervento del legislatore in materia di intercettazioni, per lo più definito «inopportuno». Il procuratore Spataro ha raccomandato di «attuare piuttosto le procedure esistenti», aggiungendo che «non è possibile che sia il legislatore a disciplinare la rilevanza delle intercettazioni». Ha aggiunto poi che «Deve essere chiaro

«Guarda caso, viene invocata sempre e soltanto nei processi ai cosiddetti colletti bianchi». Come dargli torto? Il procuratore Borrelli ha ricordato che il diritto dei difensori all'accesso a tutte le intercettazioni è incomprimibile. aggiunto inoltre che il meccanismo esistente «soddisfa tutti gli interessi in gioco». E allora perché cambiarlo? Lo stesso procuratore Pignatone ha ricordato che la «pubblicazione di intercettazioni prima del deposito è un fatto estremamente raro». Tornando alla politica, perfino Matteo Renzi ha dichiarato in più occasioni: «Non metteremo mano alle riforme delle intercettazioni». Ricordo qualche titolo di giornale per rinfrescare la memoria, «la Repubblica»: «Mano tesa di Renzi ai PM: non tocco le intercettazioni»; «Corriere della Sera»: «Intercettazioni, non si cambia»; «Il Messaggero»: «Renzi: non tocco le intercettazioni»; «il Giornale»: «Renzi si rimangia la riforma delle intercettazioni»; «l'Unità»: «Renzi ai PM: "Nessuna modifica alle intercettazioni"»; «Libero»: «Renzi: "Non toccherò le intercettazioni"». E, infatti, siamo qui a discutere l'esatto contrario di quanto affermato dal Presidente del Consiglio. Certo, sappiamo tutti qui dentro che Renzi è un mentitore seriale e compulsivo. Ma almeno mi sia data l'occasione di ricordarlo una volta ancora ai cittadini. Personalmente, sulle intercettazioni, io la penso nel seguente modo: «Sulle intercettazioni non possiamo andare contro la Corte di giustizia europea, che pone il diritto di cronaca prima di tutto, anche prima del diritto alla *privacy* - in particolare ma non solo - dei politici. A nessuno il dottore ha ordinato di fare politica e chi la fa, la deve fare anche per dare l'esempio. Il politico rappresenta le istituzioni e quindi non esistono suoi comportamenti privati che non incidano sulla credibilità pubblica». Ecco, io la penso così, ma quelle appena lette non sono parole mie. Sono dichiarazioni del numero due del Partito Democratico, Debora Serracchiani. E se le dichiarazioni di Renzi e della Serracchiani per voi del PD non fanno testo, vorrei ricordarvi allora le parole del ministro Orlando sulle intercettazioni, pronunciate quando ancora era responsabile giustizia del PD: «Con «Con la scusa della *privacy*, Berlusconi» - allora - «punta a bloccare la libertà di informazione (...)». Mi viene da dubitare che l'Orlando di allora sia lo stesso di adesso. Perfino la minoranza del PD, con Bersani, ebbe a dichiarare sulle intercettazioni: «Moody's ci declassa e noi parliamo di intercettazioni. Questo è un Governo che pensa solo agli affari suoi». Bersani non poteva essere miglior profeta in patria. Eravamo nel 2011 e si riferiva, evidentemente, al Governo Berlusconi. Non poteva sapere che Renzi avrebbe percorso la stessa identica strada cinque anni dopo. Se sia Bersani che Serracchiani non fanno parte di questo Senato, allora può essere utile ricordare cos'ha avuto modo di dichiarare sull'argomento il Capogruppo PD in Commissione giustizia sulle intercettazioni: «Eviteremo in tutti i modi che il Paese sia trascinato ancora una volta nella logica delle leggi *ad personam*. Le intercettazioni, soprattutto nel contrasto alle mafie e alla corruzione, sono uno strumento investigativo indispensabile. Ci opporremo, pertanto, a qualsiasi tentativo (...) di limitarne l'utilizzo». Era il 2013. Proprio in tema di leggi *ad personam*, questa legge non é stata forse firmata anche dal ministro dell'economia e delle finanze Padoan, la stessa persona che il ministro Guidi, intercettata, ha descritto come «messo lì dalla cricca del petrolio». E poi parliamo di leggi *ad personam*? ricapitolando, non sussistono, numeri alla mano, nessuna necessità ed esigenza di tutela della *privacy.* L'ANM, il CSM e tutti i procuratori auditi si sono dimostrati apertamente contrari e lo stesso Renzi ha rilasciato dichiarazioni su dichiarazioni contrarie nel merito. Perché dunque questa delega continua a essere imposta al Parlamento da Governo e maggioranza? Ragionevolmente, dovrebbe essere superata a causa sia delle linee guida sulle intercettazioni, che sono già state emanate da ben 19 procure, che della risoluzione del CSM sulla stessa materia. Sicuramente questa delega non viene fatta nell'interesse dei cittadini, che quotidianamente a tutto pensano meno che a essere intercettati e violati nella *privacy*. Diciamolo chiaramente: questa delega é stata pensata per una tutela della politica e dei politici dalle intercettazioni, per ridurre il pericolo che intercettazioni scomode al potere possano diventare di pubblico dominio. E ciò è ben comprensibile, se si pensa che ben tre Ministri della Repubblica hanno dovuto rassegnare le dimissioni in questa legislatura, non senza vergogna, a seguito della pubblicazione di loro intercettazioni di assoluta gravità. In qualsiasi altro Paese del mondo la politica avrebbe fatto tesoro di questi scandali per migliorare la selezione dei propri rappresentanti, soprattutto sul piano valoriale, etico. In Italia si interviene invece sulle intercettazioni, come se la causa dei numerosi scandali che si sono succeduti fosse la pubblicazione delle intercettazioni scomode alla politica, piuttosto che i gravi comportamenti da condannare che quelle stesse intercettazioni hanno reso di pubblico dominio. Questo, dunque, appare il vero obiettivo della delega: in un Paese in cui la corruzione è una primaria emergenza nazionale, al cittadino non devono arrivare informazioni che disturbino il potere e chi lo esercita. È di tutta evidenza che, poi, ci troviamo davanti a specialisti della giravolta sul bavaglio che, a seconda del tipo di intercettazioni che finiscono sui giornali, cambiano coinvolgono membri di un Governo di centrodestra, sono gli esponenti di centrodestra a proporre una stretta sulle intercettazioni e quelli di centrosinistra fingono di opporvisi. Se però le intercettazioni riguardano membri del Governo di centrosinistra, allora sono i parlamentari di centrosinistra a tentare di percorrere esattamente la stessa strada, come sta avvenendo ora. In merito alla riforma della prescrizione, arriviamo a discuterne dopo che per anni abbiamo assistito al suo oblio in un cassetto, ad assenze strategiche del relatore, al sostanziale boicottaggio da parte delle forze di maggioranza di un provvedimento divisivo, cioè in grado di incrinare la maggioranza e lo stesso Governo. Per illustrare la nostra proposta in tema di riforma della prescrizione, vorrei usare le parole del presidente della commissione di studio in tema di processo penale presso il Ministero della giustizia, Giovanni Canzio, e del professor Giorgio Spangher: «Totale condivisione della scelta della paralisi degli effetti della prescrizione con la condanna di primo grado, una tesi che ho sostenuto ripetutamente». «Il sapere che c'è uno sbocco possibile di tipo procedurale al processo, cioè il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, perverte la funzione propria del processo». Sull'argomento, il professor Spangher si esprime come segue: «L'allungamento del tempo della prescrizione e, quindi, l'impossibilità di lucrare, sul tempo del processo, un proscioglimento, porterà a un'alternativa: accedere a questi riti che hanno contenuto di condanna, con accettazione con accettazione della condanna sul materiale dell'accusa, o giocare il dibattimento sul materiale dell'accusa». ripristinerebbe nel nostro Paese un minimo Stato di diritto, reintroducendo una ragionevole certezza della pena e incentivando i riti alternativi. Ma non é solo una questione di efficacia dell'azione penale. Sospendere i termini di prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado avrebbe significative ripercussioni sulla stessa durata dei processi. Come dice Davigo: «Se vogliamo far diventare una cosa seria l'amministrazione della giustizia, dobbiamo ridurre il numero dei procedimenti e, soprattutto, il numero di impugnazioni meramente di impugnazioni meramente dilatorie sperando che il fatto si prescriva o, comunque, manifestamente infondate che vengono presentate. Ne consegue che la riforma della prescrizione rappresenterebbe uno straordinario veicolo di riduzione della durata dei processi, andando a liberare i tribunali di tutti quelle impugnazioni presentate a solo fine dilatorio, in attesa e sperando nella prescrizione». Insomma, nel momento in cui si esercita l'azione penale, un sistema civile e democratico dovrebbe dire che la prescrizione non esiste più. Ricordo, in questo senso, che il presidente emerito della Cassazione Santacroce ha definito la prescrizione «un'intollerabile abdicazione dello Stato». Come dargli torto? Con 130.000 prescrizioni all'anno, abbiamo in Italia 400 processi penali prescritti al giorno. È di tutta evidenza il clima di impunità che regna nel nostro Paese. La mancata certezza della pena rende la corruzione vantaggiosa per i criminali. Corrompere, così come commettere i reati propri dei «colletti bianchi», è un'attività che non genera rischi, perché le condanne sono evitabili grazie alla prescrizione. Nella relazione dell'Unione europea sulla lotta alla corruzione si legge: «In diverse occasioni il Parlamento italiano ha approvato o ha tentato di far passare leggi *ad personam* a favore di politici imputati in procedimenti penali, anche per reati di corruzione. Ne è un esempio la legge sulla prescrizione breve, che comporta l'elevato rischio di veder estinguere procedimenti a carico di indagati incensurati». Per l'Unione europea l'attuale disciplina della prescrizione é addirittura incompatibile con il diritto dell'Unione, tanto da invitare i magistrati a disapplicarla. Così ora i reati contro l'Unione europea in Italia non si prescrivono mai, tutti gli altri quasi sempre! Basterebbe una norma di una riga, che sospenda la decorrenza della prescrizione dal rinvio a giudizio o dalla sentenza di primo grado, per risolvere il problema una volta per tutte. Ogni diversa soluzione, mediata con coloro che non hanno alcun interesse a far funzionare la giustizia nel nostro Paese, rappresenta un inaccettabile compromesso al ribasso. Si perde un'occasione storica per ridare fiducia ai cittadini nella giustizia, per riappropriarsi di quella certezza del diritto che ormai da troppi anni nel nostro Paese é solo un flebile ricordo e, non da ultimo, per rendere molto più veloci i processi, grazie al maggior impulso che ne conseguirebbe, nel percorrere i riti alternativi. Ricordo che la revisione della normativa sulla prescrizione rientra tra le raccomandazioni che il Consiglio europeo ha rivolto all'Italia nel luglio 2013 quale importante fattore per il contrasto alla corruzione. Perfino l'OCSE nel suo *report* del 2015,

maggioranza), dall'altra afferma con forza che, per incentivare lo sviluppo economico italiano, è necessaria una legge di riforma seria della prescrizione, che non si fa.

annullerebbe sostanzialmente ogni possibilità di farla franca e renderebbe molto più probabile l'apertura delle porte del carcere, soprattutto, e in particolar modo, a molti politici corrotti, a tutti i livelli. Per questo motivo non l'approverete, nonostante le dichiarazioni più volte fatte e messe a verbale anche dal vostro Capogruppo in Commissione giustizia, secondo cui la posizione ufficiale del Partito Democratico sulla prescrizione sarebbe in linea con la proposta del Movimento 5 Stelle, e nonostante le moltissime firme che, voi voi parlamentari del Partito Democratico, avete posto a disegni di legge o emendamenti che andavano esattamente nella direzione da noi auspicata. Si tratta di provvedimenti annunciati e poi imboscati, ritirati o a cui sono state tolte le firme per non indisporre Alfano, Verdini, Schifani, Formigoni o Azzollini. È il trionfo dell'ipocrisia. Non vi preoccupate, ne terranno in debito conto gli elettori alla prima elezione possibile. La riforma della prescrizione la faremo noi, non appena vi avremo mandato a casa, con buona pace di quanti, ancora adesso e anche in quest'Assemblea, credono di poterla fare sempre franca, così come stanno facendo da troppo tempo. Grazie Presidente. l'articolo 111 della Costituzione statuisce: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

supponiamo che questo sia. Abbiamo subito un sintomo che ci dice che probabilmente questo non avverrà, perché - contemporaneamente - ci viene proposto un aumento spropositato dei tempi della prescrizione. Se i processi si faranno più velocemente, si poteva non intervenire sulla questione della prescrizione, che era già stata toccata undici anni fa, con il risultato, tra l'altro, di una forte riduzione - che, negli anni, è diventata un dimezzamento - dei processi che cadono in prescrizione. Mi sto rifacendo a dati che ci sono stati forniti

previsione della Costituzione stabilisce che il processo deve avere una ragionevole durata? Si allungano i termini di prescrizione. I casi sono due: o si sta facendo una cosa schizofrenica (ossia si fa una cosa totalmente irrazionale),

il processo dovrebbe servire; e il processo serve perché non tutti gli imputati sono colpevoli per definizione. Altrimenti, se fossero già colpevoli a che servirebbe il processo?

La giustizia può sbagliare, tant'è vero che la giustizia prevede tre gradi di giudizio. Sappiamo che il terzo non è uguale al secondo ma, tal proposito, mi viene qui in mente un'analogia: si dice che Camera e Senato fanno lo stesso lavoro; bene, anche il tribunale di primo grado e quello di secondo grado fanno lo stesso lavoro, eppure,

Ecco perché esiste il termine di prescrizione. Ed esiste anche in nome, e anche prima, di quella norma costituzionale secondo cui il processo avviene su un piede di parità. Non può esserci parità tra l'imputato e lo Stato che lo accusa: infatti il procuratore che accusa si chiama procuratore nientemeno che «della Repubblica». Credo che tutti noi che abbiamo visto qualche telefilm giudiziario siamo rimasti colpiti dalla formula con cui inizia un processo negli Stati Uniti (da noi no, perché non lo si dice, ma è così). si dice: «lo Stato del Texas contro il signor Smith». Accidenti, lo scontro è impari: il povero signor Smith è da solo, magari è povero, magari ha un avvocato che non è un granché, mentre lo Stato del Texas è grande e potente. potente. La stessa cosa accade da noi: è la Repubblica, di cui l'accusatore per l'appunto è il procuratore, contro il signor Rossi. Il signor Rossi deve avere il diritto di difendersi, la Repubblica ha diritto a condannare il signor Rossi se quest'ultimo viene trovato colpevole, ma ci deve essere un piede di parità. Non c'è parità in una partita se una parte ha in mano la possibilità di stabilire quando la partita finisce. Non ci sarebbe parità in un qualsiasi incontro sportivo in cui una parte avesse la possibilità di stabilire quanto dura questo incontro. allora non solo la possibilità che, in buona fede, un innocente venga tenuto anni e anni "sotto schiaffo", in una situazione di cui dobbiamo considerare non soltanto gli aspetti psicologici

però eri innocente? Ma in trent'anni questa persona ha avuto la vita distrutta. E bastano molto, molto meno di trent'anni perché una persona accusata veda distrutta la propria vita: famiglie distrutte, prestigio professionale azzerato, perdita del lavoro e dei propri redditi. Ecco perché è bene che ci siano dei limiti. Aggiungete che non è impossibile che ci sia un certo arbitrio da parte di alcuni magistrati; certamente una minoranza, ma può succedere.

che un giudice che non sia in grado di portare alla condanna una persona verso la quale ha ostilità, faccia la cosa peggiore: pur conoscendo la sua innocenza,

Del resto, ci sono organismi che sono lì per giudicare eventuali colpe di magistrati che non facciano bene il proprio lavoro (poi quanto approfonditamente lo facciano è un'altra faccenda), quindi può succedere. Ci deve essere allora un limite. Il magistrato può avere un'ostilità, magari anche giustificata. quel magistrato che voleva mettere in carcere Al Capone negli Stati Uniti, non riuscendo a metterlo in carcere per i tanti efferati delitti, omicidi e quant'altro aveva compiuto, riuscì a farlo per evasione fiscale. Sicuramente aveva un'ostilità nei confronti di questa persona, ma ha avuto un tempo limitato entro il quale poter mettere e poi ricordiamoci che la prescrizione facilita e incoraggia l'allungamento dei processi, in generale, lasciando stare casi di malanimo o addirittura di parzialità del giudice. Sappiamo benissimo dalla cronaca e molto bene molto bene da quello che gli stessi magistrati dicono, e cioè che cercando lodevolmente di non mandare in prescrizione dei processi, quelli che sono prossimi alla prescrizione li si accelerano. Qui invece cosa facciamo? Allunghiamo la prescrizione come a dire che per tempo. Stiamo facendo una cosa razionale riducendo i tempi dei processi e poi allungando la prescrizione? Direi proprio di no. Accanto a questo, ci sono alcuni altri problemi nel disegno di legge di cui approfonditamente ha parlato il senatore Caliendo. A me colpiscono due aspetti: il riordino dell'ordinamento penitenziario e il riordino della disciplina che riguarda le intercettazioni telefoniche. Il senatore Cappelletti che mi ha preceduto ha citato le numerose numerose occasioni in cui il Presidente del Consiglio, e non solo lui (anche il Ministro della giustizia), ha detto che non avrebbe modificato le prescrizioni. Stranamente, anche in quel caso, come in quasi tutti gli altri, il Presidente del Consiglio si è poi smentito

ora ha deciso di farlo, per di più per delega, cioè affidando a sé praticamente il compito di scrivere la norma. Ebbene, mettendolo insieme all'articolo principale che c'è oggi sul nuovo quotidiano «La Verità», riguardante certe intercettazioni che riguardano la famiglia del Presidente del Consiglio, mi è venuta in mente la celebre frase di quell'attore genovese che, essendogli stato annunciato che un tale,

con il provvedimento che stiamo discutendo oggi mettiamo un altro tassello importante a quella necessaria riforma della macchina della giustizia nel nostro Paese, che rappresenta oggi una delle sfide più impegnative per questo Governo, per questa maggioranza e per il Paese tutto. Sappiamo bene come una serie di malfunzionamenti che riguardano proprio la macchina della giustizia siano profondamente connessi con una serie di malfunzionamenti del sistema del sistema Italia, che non riguardano solo il tema della maggiore tutela dei diritti dei cittadini, ma lo stesso funzionamento del nostro sistema. Riguardano la capacità dell'Italia di essere attrattiva rispetto

superando quell'ampia serie di mali che - dalla corruzione alla più generale mancanza di regole, all'incapacità di vedere nel sistema giudiziario un effettivo luogo di tutela dei diritti delle persona - mette in crisi o rappresenta un limite importante rispetto al fatto che l'Italia sia un Paese considerabile, secondo criteri nuovi, moderni aggiornati, esigenti, uno Stato di diritto in piena regola. Mi soffermo brevemente sulla questione

Sulla prescrizione, insieme alla senatrice Ricchiuti e al senatore Tocci, avevo presentato una proposta che indicava un modello differente rispetto a quello che è stato adottato da questo provvedimento. una proposta che, facendo proprio un ragionamento che in dottrina trova forti sostegni e condivisioni, andava a distinguere due elementi, elementi, che noi con un termine generale chiamiamo prescrizione, ma che in realtà sono molto diversi tra di loro. Mi riferisco cioè a quella fase, a quel tempo puramente cronologico che scorre dalla commissione del reato fino all'avvio del procedimento

dall'altra parte, trova però un suo limite nell'esigenza del cittadino di non vedersi addosso la spada di Damocle di un procedimento che dura all'infinito; vi è poi un altro tempo che a mio avviso viene impropriamente considerato un tutt'uno con il primo ed è quello del processo. Quella proposta indicava una strada, cioè la distinzione netta tra queste due fasi: un tempo di prescrizione ma che si interrompeva definitivamente nel momento dell'avvio del procedimento, accompagnando però questo con un secondo tempo della prescrizione, cioè non più legato allo scorrere cronologico del tempo, ma ai diversi passaggi del processo. del processo. In questo secondo tempo il superamento della ragionevole durata di ogni passaggio avrebbe potuto comportare un abbassamento della sanzione prevista, fino al suo annullamento complessivo per il cittadino che si vedesse costretto dalla lunghezza dei tempi del processo a un'attesa spropositata rispetto al suo diritto a vedersi processare in tempi brevi.

quelli la cui prescrizione frequente (penso ai reati dei colletti bianchi) rappresenta una fonte di scandalo motivato per l'opinione pubblica del nostro Paese. Rispetto al tema della prescrizione, insieme ad altri ad altri senatori ho sottoscritto un paio di proposte di emendamento che mi auguro possano essere tenute in considerazione da quest'Assemblea e che riguardano alcuni casi specifici.

in cui è in gioco il bene della vita e in situazioni in cui anche a lunga distanza di tempo è possibile individuare i responsabili del reato (solo in queste situazioni) tali emendamenti propongono il termine della prescrizione decorra dal momento in cui la notizia di reato venga acquisita o pervenga al pubblico ministero.

tema della riforma dell'ordinamento penitenziario, che nel provvedimento oggi in esame è contenuto nel Titolo IV. Voglio salutare positivamente una parte: mi riferisco in modo specifico all'articolo 36, contenente i principi di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, che a mio giudizio tiene conto positivamente, in modo anche articolato, di quel processo importante che è stato rappresentato dagli Stati generali dell'esecuzione penale, i cui lavori hanno avuto luogo nei mesi scorsi e che hanno visto all'opera e al confronto le migliori energie che nel nostro Paese, a titolo diverso, si occupano dell'ordinamento penitenziario e hanno ispirato una serie di misure che in una concretizzazione. Di questa parte degli elementi indicati nella delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario voglio sottolineare alcuni aspetti,

abbiamo già attivato una serie misure orientate a ridurre il sovraffollamento carcerario; lo abbiamo fatto sulla spinta di una sentenza a noi negativa, una sanzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ci aveva condannati per il sovraffollamento delle nostre carceri. Ma questa azione può continuare anche oggi che un sovraffollamento esiste ma è molto limitato nei numeri rispetto a quanto accadeva solo un paio di anni fa. Questa strada ci può condurre a ragionare in maniera

la strada privilegiata per il reinserimento sociale, per la riduzione della recidiva e per il superamento di una situazione di criminalità che, per uno Stato democratico e di diritto, devono essere

la recidiva diminuisca laddove si ha la possibilità di accedere a sanzioni alternative alla detenzione. di norme che facilitino il ricorso alle misure alternative; bene l'eliminazione di quegli automatismi impeditivi della possibilità di usufruire impeditivi della possibilità di usufruire di misure alternative al carcere e bene anche il superamento, a determinate condizioni e fatti salvi alcuni particolari delitti, delitti, della preclusione dei benefici a chi è condannato alla pena dell'ergastolo. Voglio sottolineare uno dei

A questo proposito, mi auguro - e ho presentato un emendamento in questo senso - che ci possa essere da parte di quest'Assemblea un'attenzione per una maggiore articolazione di questo punto,

la sanzione della detenzione non sia accompagnata da un processo di abbrutimento e di sterilizzazione delle relazioni affettive e familiari delle persone detenute. Da un lato c'è l'obiettivo, per l'appunto, di un corretto, salutare e positivo reinserimento sociale, anche dal punto di vista del proprio nucleo familiare e della propria rete affettiva, da parte di chi sia condannato ad una detenzione

di terzi o di incontro con i familiari in apposite aree e la previsione di un incremento del numero di minuti settimanali dedicati alla possibilità di telefonare casa o una sostituzione di quei colloqui, che spesso chi ha i familiari lontani non può fare, con ulteriore minuti di colloquio telefonico. Sarebbero tutte misure che andrebbero nella direzione di rendere il carcere un luogo che effettivamente prepara i detenuti ad un reinserimento sociale e non un luogo di produzione di recidiva. Voglio ricordare ancora alcune altre misure, che sono state inserite nel provvedimento a seguito dell'accoglimento in Commissione di emendamenti presentati dal mio Gruppo. Mi riferisco, ad esempio, a norme che considerino i bisogni specifici delle donne detenute. Oggi il fatto che le donne rappresentano, dal punto di vista percentuale, una una quantità molto piccola rispetto al totale della popolazione carceraria fa sì che il sistema detentivo sia a misura d'uomo e che non si prendano in considerazione in maniera adeguata le specificità delle donne nel periodo della detenzione. Una cosa

anche per le donne incinte o madri di bambini molto piccoli detenute in situazione di carcerazione provvisoria, valga quel principio inderogabile che il nostro ordinamento prevede per le donne incinte o con bambini molto piccoli condannate in via definitiva, cioè la totale incompatibilità con la situazione detentiva. Oggi noi viviamo il paradosso per cui una donna condannata con un bambino piccolo può usufruire di situazioni alternative alla detenzione, invece una donna che sia in carcere in attesa di giudizio può essere sottoposta a un giudizio discrezionale da parte del giudice. Il principio di delega, che questo provvedimento ha già fatto suo tramite un emendamento approvato in Commissione, prevede per l'appunto che anche all'imputata sottoposta a misura cautelare si garantisca quella stessa situazione di sospensione della detenzione fino al momento in cui il figlio o i figli abbiano compiuto il primo anno di età. C'è poi un altro punto che riguarda sempre i diritti delle persone detenute: mi riferisco al tema della libertà di culto. non esiste, all'interno delle nostre carceri, un principio di riconoscimento paritario del diritto alla libertà di religione per chi professa religioni differenti. Per chi professi religioni diverse da quella cattolica c'è spesso una difficoltà totale rispetto alla possibilità di vivere la propria religiosità all'interno dei luoghi di detenzione. che, per quanto possibile in una situazione di parità, si garantisca a tutti la possibilità di poter esprimere la propria libertà la propria libertà di culto. Ancora, sottolineo un altro aspetto contenuto nel provvedimento: il fatto che si superi quell'incongruenza per cui spesso le misure accessorie - penso per esempio all'interdizione dai pubblici uffici o a alla perdita del diritto di voto - abbiano una durata superiore rispetto alla durata della pena principale. Questo è un *vulnus* che va riparato - e questo provvedimento se ne fa carico - per un motivo molto semplice: gravare su una persona che abbia terminato il periodo di detenzione con un impedimento a un pieno reinserimento sociale significa ribaltare quella logica che vuole che lo Stato si faccia carico di accompagnare (e questo succede purtroppo ancora oggi in maniera assolutamente insufficiente) la persona che abbia scontato la sua pena e che abbia pagato il suo debito con la giustizia verso un reinserimento positivo

residenze sanitarie che abbiamo varato nel momento in cui sono state superate quelle strutture desuete che erano gli OPG, ossia gli ospedali psichiatrici giudiziari. Ho sottoscritto

ripristina quel principio per cui all'interno delle residenze sanitarie, le REMS, destinate a chi si trova in una situazione di instabilità psichica, abbiano accesso solo quelle persone di cui in maniera definitiva sia stato accertato lo stato e che scontino una pena definitiva, lasciando invece che le persone il cui stato

avendo un disagio psichico, a dover scontare una pena all'interno di un istituto di detenzione, trova un suo fondamento in un altro principio principio di delega che è contenuto nella lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 36, laddove si parla di

un impegno specifico affinché effettivamente, all'interno di tali istituti, ci sia quel potenziamento dell'assistenza psichiatrica che, in conseguenza del riordino della medicina penitenziaria, previsto dal decreto legislativo n. 230 del 1999, faccia sì che anche l'istituto penitenziario possa assolvere questo obbligo di legge nella maniera più proficua possibile.

si parla di riforma e quindi ci si aspetta naturalmente un provvedimento globale, complessivo: un provvedimento che, in effetti, aveva in origine l'ambizione di risolvere tutta una serie di problemi che sono sotto gli occhi di tutti e che affliggono la giustizia penale. Ora ci si ritrova davanti a un provvedimento che, in ragione di un legittimo nonché positivo lavoro in Commissione,

i problemi della giustizia penale sono stati oggetto di numerose discussioni all'interno di questa Assemblea. Sicuramente il disegno di legge dispone soprattutto sul versante processuale, scendendo nel dettaglio. Domandiamoci invece quanto del funzionamento della giustizia, più che dipendere dall'intervento del legislatore, dipenda dall'attività dell'Esecutivo e cioè dal Ministero della giustizia e da tutte le sue articolazioni,

si aprono anche fronti di grande contraddizione. Da un lato c'è l'innalzamento delle pene per dei reati contro il patrimonio e dall'altro ci sono deleghe per favorire enormemente le misure alternative alla detenzione.

ripensamento della giustizia ci sia un continuo, lento e gocciolante interesse e un'attenzione per i reati contro il patrimonio, pubblico e privato, e parallelamente ci sia una continua diminuzione dell'attenzione per i reati nei confronti della persona. Credo che ciò non aiuti una affermazione, che poi passa anche per fenomeni di osmosi culturale, e un'adeguata realizzazione della cultura del rispetto delle persone e anche, in un secondo momento, del rispetto del patrimonio e di tutto quello che è il terreno del pubblico. Le modifiche sono inoltre eterogenee anche rispetto alla loro stessa formulazione. Da un lato abbiamo degli interventi molto specifici, dall'altro dall'altro abbiamo ampie deleghe. Negli interventi specifici e nelle deleghe c'è un principio più e più volte esibito, anche a mezzo stampa e durante i lavori in Commissione.

non hanno accolto nulla delle osservazioni fatte. Devo dire che il ministro Orlando si è presentato, ha accolto, ha ragionato e ha discusso e questo sicuramente ha dato dignità ai lavori della Commissione, cosa che altri suoi colleghi non fanno.

grado. Il messaggio che voglio dare, per quanto riguarda la prescrizione, tema che ha molto appassionato, è che comunque il problema si risolverebbe se i tribunali fossero messi nella condizione di lavorare con tutte le risorse disponibili

voleva proporre e che, forse, non ha osato proporre. Quando ho chiesto che si affrontasse in modo contestuale il nodo della cura, ma anche della pericolosità, è è nata la discussione. Ora, i toni apocalittici, che usa la senatrice Dirindin quando considera il testo approvato, sono la dimostrazione del fatto che, in realtà, le articolazioni sanitarie, cui faceva appello anche il senatore Lo Giudice, sono totalmente inadeguate. Il fatto che oggi si voglia creare una platea

«nonché» gli altri «qualora» negli istituti penitenziari non siano state attivate quelle articolazioni che per legge dovrebbero esserci. si abbia paura di questa formulazione è la dimostrazione che si sa perfettamente che il sistema sanitario e il sistema penitenziario certamente non sono nell'immediato - e, forse, anche non nell'immediato - nella condizione di poter dare delle risposte vere a quella popolazione

mi sembra venga totalmente sottovalutato, ossia che il problema della giustizia riguarda i cittadini. In uno Stato di diritto e democratico un cittadino

a cui deve sottostare per uno, due, cinque, dieci, trenta o quarant'anni, senza che lo Stato abbia la compiacenza di dirgli se è innocente o colpevole. Mi è già capitato di sottolineare un altro

si insisteva nel rilanciare, più le leggi non venivano attuate. Stiamo oggi rimettendo mano, per la terza o quarta volta in quattro anni, a norme penali.

Come ho detto e continuo a ripetere, senza citare casi da me già riportati, più l'arresto è ingiustificato, più l'errore del magistrato è eclatante, più quel processo non si farà. E questo non perché chi è finito in galera non vuole più che si tenga il

Sto parlando di anni e anni: tre anni, quattro anni, cinque anni, sei anni prima ancora del processo di primo grado. Ammesso, poi, che chi è stato arrestato si ricordi ancora le ragioni le ragioni del fatto. Richiamo i casi dell'Aquila o di Terni, ma potrei citare decine di casi di questo genere. Quindi, abbiamo alzato le pene in maniera tale che si parta con l'arresto.

oggi si va da sei anni a sette anni e sei mesi, così come era prima della legge n. 69 del 2015. Con queste modifiche si porta il

come il *requiem*: non ci deve essere un limite che lo Stato si pone per perseguire un cittadino. Il cittadino teoricamente può stare sotto processo tutta la vita.

fiducia, farà passare un testo sul quale c'è un piccolo problema politico che vorrei sottolineare. Ho sentito i colleghi di AL-A dire che non voteranno la fiducia.

l'aumento della prescrizione era già arrivato al limite massimo di sopportazione per la lesione di principi costituzionali e per una questione di moralità pubblica, di atteggiamento dello Stato verso i cittadini. Mi sembra di capire che questo giuramento o promessa solenne di fare una battaglia all'ultimo sangue per evitare che questo accada, come al solito finirà con Area Popolare che cede con fermezza.

far passare questa cosa incredibile verranno da quel partito che ha sempre sostenuto non dico posizioni garantiste, ma vogliamo dire posizioni di buon senso?

di omicidi o di simili reati, è evidente che non c'è prescrizione e quindi la pretesa punitiva dello Stato deve continuare nel tempo, ma per le cose di cui stiamo parlando (l'induzione, la corruzione per un atto proprio del pubblico ufficiale), pensate che dieci o quindici anni dopo sia possibile andare a ricostruire

comportarsi nella stessa maniera. Ho sempre considerato un sistema barbaro ed incivile quello di eliminare dalla vita politica e amministrativa una persona semplicemente per il fatto che è stata iscritta nel registro degli indagati, cosa che non vuole dire assolutamente nulla.

a Casson, la prescrizione perpetua; AL-A e Area Popolare fino a ieri non la volevano; il risultato è che politicamente, se passerà questa fiducia, significa che qualcuno ha ceduto completamente sulle sue questioni di principio, visto che quella che stiamo sollevando - continueremo a farlo in maniera decisa - è una questione di grande principio, da cui deriva deriva la civiltà giuridica di un Paese. Questo provvedimento non ci fa fare un passo avanti nella civiltà giuridica, ma un passo drammaticamente all'indietro, lasciando il cittadino colpevole o innocente - e tantissime volte innocente - in balia delle istituzioni.

i 40 articoli dei quali si compone il provvedimento all'esame dell'Assemblea recano significative modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale. Un provvedimento che si inserisce nella prospettiva riformistica portata avanti in questi ultimi tre anni, anche nel fondamentale settore della giustizia penale. La nostra idea di riforme ha come obiettivo la piena attuazione del modello di giurisdizione e del sistema di garanzie contenuti nella nostra Carta fondamentale. Le nostre proposte riformatrici mirano a realizzare pienamente l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Per questo non possono restare mere disposizioni non solo l'articolo 3, ma anche l'insieme delle norme costituzionali che regolano il funzionamento della giustizia: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva; il diritto alla ragionevole durata del processo; il diritto alla difesa garantito anche ai non abbienti e infine la finalità riabilitativa della pena. Attuare la Costituzione significa, prima di tutto, rimuovere le vere emergenze che caratterizzano il servizio giustizia e che impediscono l'esercizio di diritti fondamentali. Significa garantire un giusto processo che, per tempi e modalità, riduca il rischio di discriminazioni originate da differenze sociali di razza o di sesso, sia per chi è imputato sia per chi fa valere un suo diritto o è parte offesa o vittima di un reato. Per questo, infine, è necessario adeguare l'ordinamento in modo funzionale al pieno perseguimento di questi obiettivi, anche valorizzando e qualificando l'attività e la professionalità di tutti gli operatori del servizio giustizia. In particolare, il provvedimento in esame, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, interviene sulla disciplina di alcuni reati: tra gli altri, i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina, inasprendone il quadro sanzionatorio. In particolare, l'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter*, inasprendone il quadro sanzionatorio. È opportuno ricordare in proposito che, nel corso dell'attuale legislatura, la legge del 17 aprile 2014, n. 62, ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione, oltre che di denaro, anche di altre utilità. Sotto il secondo profilo, ha ridotto invece la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter*, con la pena della reclusione da quattro a Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da sei a dodici anni. Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: rispettivamente del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), del furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene ed escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze. mi accingo a svolgere riguarda la necessità di dare un quadro organico al sistema sanzionatorio relativo

elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). La disposizione, inoltre, inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto, di cui all'articolo 625 (vedi articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti. L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500. L'articolo 6 L'articolo 6 interviene sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro nel massimo). La disposizione inasprisce inoltre anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con un'altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (cioè le aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione (altro capitolo importante), con particolare riguardo ai reati di corruzione. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. A questo proposito l'articolo 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega, inoltre, l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni - dall'ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona;

prevedendo che sia il pm a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a rimodulare altresì i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo, poi, delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare. Infine, l'articolo 14 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge. Il testo contiene poi importanti modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi in materia d'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; sulla disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; sulla disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; per la semplificazione delle impugnazioni e per la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo, il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici, e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri. In particolare si prevedono per la riforma dell'ordinamento penitenziario le seguenti misure: anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari; la previsione di attività di giustizia riparativa; l'incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario che esterno, nonché di attività di volontariato; revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria (anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi e al riconoscimento del diritto all'affettività; interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri; stranieri; l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto la tutela di beni di rilevanza costituzionale (i beni della salute individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico e di mercato). Parliamo anche della previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica; interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri; di una revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli, al reinserimento sociale del condannato e all'esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale; revisione, infine, delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi. La delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione e ai contatti con la società esterna in funzione del reinserimento sociale. signor Presidente, che questa esposizione abbia dato contezza della complessità di questo provvedimento, ma anche della volontà precisa di andare a riformare delle parti del nostro ordinamento che sono assolutamente importanti e decisive per dare efficacia reale allo stesso e soprattutto per garantire la possibilità di agire, attraverso il processo, in modo tale da dare certezza alle pene, ma anche una reale possibilità di recupero e di riabilitazione

credo che rappresenti un fatto veramente significativo. Poi sicuramente la discussione in Assemblea metterà a fuoco alcuni elementi che meritano un ulteriore approfondimento e probabilmente portano con sé la necessità di svolgere riflessioni

indipendentemente dal ruolo che ricoprono nel momento in cui sono sottoposti ad un procedimento giudiziario.

due tecnici italiani e un canadese operanti in blocco per la ditta Conicos, società di Cuneo attiva nell'ambito della manutenzione del locale aeroporto. La città è sotto il controllo del governo di unità nazionale di Tripoli riconosciuto a livello internazionale. I tre sono stati probabilmente rapiti da soggetti noti alle autorità locali per avere in passato effettuato imboscate e rapine, secondo quanto riferisce il portavoce della municipalità di Ghat. Signor Presidente, auspico che il Governo segua con tutta l'attenzione necessaria questa ennesima situazione di crisi e non risparmi alcuna iniziativa per permettere, in particolare ai due italiani, provenienti l'uno da Cuneo e l'altro da Belluno, di riabbracciare a breve i propri familiari. Mi auguro allo stesso tempo che i servizi del Ministero degli affari esteri e di Palazzo Chigi stiano vicini alle famiglie in questo momento di profonda apprensione per la sorte dei propri congiunti. Vi sarà successivamente il tempo per approfondire le motivazioni e le valutazioni che solo due giorni prima, secondo notizie di stampa, hanno portato alla decisione di togliere la scorta ai tecnici. Ora è il momento di agire per riportare a casa indenni i nostri concittadini. La ringrazio anche per avere richiamato l'attenzione del Senato e delle istituzioni tutte su questa drammatica emergenza, che immagino vedrà impegnate con solerzia tutte le autorità competenti con l'efficacia che il caso impone.